Presidente, intervengo per denunciare un fatto molto grave che ha leso la dignità del Senato della Repubblica.

attraverso un compenso pattuito di 3.500 euro mensili netti, per quindici mensilità, per l'intero periodo residuo della legislatura. A questo punto, presidente Marini, per la dignità di questo ramo del Parlamento, la invito a verificare, in relazione ai suoi poteri e doveri, se il senatore Luigi Malabarba si sia dimesso a seguito di un accordo economico con il suo Capogruppo, che avrebbe utilizzato per liquidarlo i contributi versati dall'amministrazione del Senato della Repubblica al Gruppo di Rifondazione Comunista.

Concludo, signor Presidente, sottolineando che, se i fatti denunciati rispondessero invece al vero, sarebbero di una gravità inaudita. In tal caso, i colleghi di Rifondazione Comunista coinvolti nella vicenda, oltre a dover subire le conseguenze penali ed amministrative per i reati commessi (si parla di 110.000 euro versati in contanti per sanare questa vertenza), dovranno essere duramente censurati dal Senato per avere leso la dignità di questo ramo del Parlamento. Recentemente, per voti di fiducia si è parlato di vendita di voti. Credo che qui siamo ai saldi di fine stagione, ovviamente politica!

la votazione per l'elezione di due senatori Segretari. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2-*bis*, del Regolamento, i Gruppi Misto e Democrazia Cristiana-Partito repubblicano per l'Autonomia hanno avanzato la richiesta di procedere all'elezione di altri senatori Segretari. Tale richiesta è stata accolta dal Consiglio di Presidenza dopo una procedura molto approfondita, che abbiamo affidato anche alla Giunta per il Regolamento. Procediamo dunque alla votazione. In base a quanto stabilito dal comma 2-*ter* dell'articolo 5 del Regolamento, ciascun senatore scriverà sulla propria scheda un solo nominativo. Risulteranno eletti coloro che, essendo iscritti ai Gruppi richiedenti, otterranno il maggior numero di voti, limitatamente ad un senatore per Gruppo. Dopo l'effettuazione della chiama le urne resteranno aperte fino alle ore 12,30, mentre l'Assemblea proseguirà nell'esame del successivo punto all'ordine del giorno. I senatori, chiamati in ordine alfabetico, passeranno sotto il banco della Presidenza e deporranno la scheda nell'urna predisposta.

reca: «Comunicazioni del Governo sulla liberazione del giornalista Daniele Mastrogiacomo». Dopo l'intervento del rappresentante del Governo, ciascun Gruppo ha a disposizione dieci minuti; quindici il Gruppo Misto.

Signor Presidente, onorevoli senatori, il 5 marzo il quotidiano «la Repubblica» ha avvisato l'Unità di crisi del Ministero degli affari esteri di aver perso i contatti, dal giorno 4 marzo, con il proprio inviato Daniele Mastrogiacomo, che dall'Afghanistan, nell'ultima conversazione telefonica con i suoi colleghi, aveva annunciato di avere in programma di recarsi nella provincia meridionale di Helmand per fare un'intervista ad un capo dei talebani. Trattandosi di una zona ad elevato rischio - nella quale era in fase di avvio un'importante operazione militare - il Ministero degli esteri ha immediatamente allertato ogni possibile canale, anche attraverso l'ambasciata a Kabul, per acquisire elementi certi sulle circostanze che hanno determinato il mancato contatto di Mastrogiacomo con la redazione di «la Repubblica». Gli organi di stampa hanno in un primo tempo annunciato il sequestro di un giornalista britannico e di due accompagnatori afgani. È successivamente risultato Nell'apprendere la notizia, il Ministero degli affari esteri ha stabilito la necessaria concertazione con le altre amministrazioni dello Stato, innanzitutto con la Presidenza del Consiglio, il Ministero della difesa ed i Servizi di informazione. Uno stretto raccordo operativo è stato attivato anche con il quotidiano «la Repubblica» e con i familiari, che sono stati puntualmente aggiornati di tutti gli sviluppi della vicenda. A livello internazionale, il Governo ha in primo luogo richiesto, ai massimi livelli, la collaborazione del Governo afghano, per assicurare una rapida liberazione di Mastrogiacomo, mettendo in atto tutte le possibili misure necessarie per assicurare in ogni caso l'incolumità dell'ostaggio. Il Governo afgano ha assicurato piena collaborazione in tutto il periodo che ha condotto alla liberazione dell'ostaggio. Il Governo ha anche chiesto la collaborazione dei Governi della coalizione internazionale in Afghanistan, ed in particolare di quello americano e di quello inglese, disponendo quest'ultimo di truppe attive nell'area. Agli alleati le cui truppe erano attive nell'area è stato richiesto di evitare azioni di forza. A fronte del proliferare di notizie di stampa spesso discordanti e contraddittorie, il Ministero degli affari esteri ha escluso l'avvio di trattative fino a quando non fossero emerse prove che l'ostaggio fosse in vita ed ha chiesto agli organi di informazione di astenersi dal diramare notizie non controllate, accertate nel merito e nell'attendibilità delle fonti. Nello stesso tempo, il Governo ha continuato a seguire con attenzione tutti possibili canali di trattativa ritenuti attendibili. Il 10 marzo il Governo è venuto in possesso di elementi che hanno permesso di accertare l'esistenza in vita dell'ostaggio attraverso un canale individuato da «la Repubblica» per il tramite di un suo giornalista *free-lance* a Kandahar. Parallelamente, Gino Strada, fondatore di Emergency, ha confermato che questa ONG avrebbe potuto mettere a disposizione un canale di trattativa. Il 13 marzo è stato consegnato dai rapitori attraverso emissari di Emergency un video, risalente a due giorni prima, nel quale venivano mostrati in vita Mastrogiacomo e l'interprete afghano Ajmal Nashkabandi. Il 15 marzo l'agenzia di stampa afghana Pajhwok ha diffuso un messaggio audio in cui Mastrogiacomo confermava l'esistenza di un *ultimatum*. Successivamente la stessa agenzia ha diffuso la notizia dell'uccisione dell'autista Sayed Agha. Parallelamente sono stati mantenuti contatti con il canale individuato da «la Repubblica» che, nel corso della trattativa, ha dimostrato di avere indizi convergenti con quelli trasmessi da Emergency. Tuttavia, si è sempre privilegiato il canale aperto da Emergency perché ritenuto in grado di avere diretto accesso ai rapitori per individuare le rivendicazioni avanzate e per verificare la disponibilità ad una trattativa. Numerosi interventi istituzionali, ai massimi livelli, si sono susseguiti per chiedere al Governo afgano di mettere in atto ogni misura volta a garantire il rilascio degli ostaggi in condizioni di incolumità. Grazie a questi interventi, il 18 marzo, il Ministero degli affari esteri ha potuto confermare che tutte le condizioni poste per la liberazione erano state realizzate e ha chiesto il silenzio stampa. Al riguardo si conferma che il Governo afgano ha concesso la libertà di cinque talebani detenuti presso le carceri di Kabul affidandoli ad Emergency, il cui operato è stato determinante anche e soprattutto nella fase di scambio degli ostaggi e nel condurre in zona sicura Daniele Mastrogiacomo. Il 19 marzo il giornalista è stato rilasciato e portato all'ospedale di Emergency di Lashkargah da dove è rientrato in Italia il giorno successivo. L'azione del Governo è stata sostenuta per l'intero corso della crisi da tutte le nostre istituzioni, anche sul terreno, con la consueta discrezione, professionalità ed efficacia.

Non è stato possibile avere conferma della consegna del corpo dell'autista Sayed Agha, barbaramente assassinato. Ai suoi familiari il Ministro degli affari esteri ha manifestato la vicinanza, la commossa partecipazione del Governo e del popolo italiano.

Signor Presidente, ci troviamo qui a chiedere al Governo di fare pubblicamente chiarezza su tutti gli avvenimenti antecedenti e concomitanti, ma soprattutto sulle modalità e condizioni che hanno portato alla scarcerazione del giornalista Daniele Mastrogiacomo, vittima dei terroristi talebani e dei loro famigerati metodi criminali. Riteniamo che chiarezza in una vicenda come questa sia assolutamente necessaria, soprattutto perché temiamo - e a buona ragione - che le azioni poste in essere dal Governo per raggiungere tale fine possano costituire un pericolosissimo precedente, che temiamo nuocerà a molti nostri connazionali, i quali verrebbero a trovarsi loro malgrado a divenire merce preziosa di scambio nelle mani di uomini spietati e senza scrupoli che agiscono in nome di una insana follia di vendetta contro il mondo occidentale. Una dimostrazione lampante ci è pervenuta proprio dall'evolversi delle richieste avanzate nei lunghi giorni del sequestro, che hanno costretto a premere per concedere la libertà, dopo un balletto di numeri, a ben cinque pericolosi criminali. Naturalmente siamo più che sollevati dall'esito positivo che ha avuto questa vicenda, ma non possiamo tuttavia tacere le molteplici perplessità che ci affliggono, soprattutto alla luce delle recenti affermazioni di un autorevole membro di questa maggioranza, il quale auspica la formazione di un tavolo di pace (e fin qui andrebbe bene) a cui dovrebbero sedere i portatori di morte e di barbarie (e questo non va bene). Molti di noi speravano che le insensate parole dette dall'onorevole Fassino nei caldi giorni delle trattative fossero state dettate nell'ambito di una più globale strategia diretta a conseguire l'ambita liberazione del nostro concittadino. Ma in questi giorni, successivi alla lieta notizia, abbiamo potuto constatare come invece le stesse parole fossero in realtà portatrici di una reale quanto discutibile volontà di avvicinare queste frange estreme, che del terrore hanno fatto bandiera, ad un tavolo comune con chi della pace vorrebbe essere testimone. È ancora una volta lampante come la maggioranza si sia fatta portatrice di confusione e contraddittorietà, ancora una volta si è scoperta divisa, ancora una volta si è trovata coinvolta in un'aspra polemica a causa di comportamenti ambigui quanto pericolosi di alcuni suoi esponenti, e tutto per conquistare una manciata di voti della sinistra estrema. «Parigi val bene una messa», signor vice Ministro. In nome della conservazione di un traballante potere si è arrivati a proporre di dare voce a chi delle parole non si è mai servito, a chi conosce solo la lingua del terrore e del sangue, a coloro i quali rinnegano la pace come concetto di pacifica convivenza in un Paese libero e democratico. Com'è possibile parlare di dialogo con chi proprio ieri si è reso ancora una volta colpevole del ferimento di un membro delle nostre truppe? Allora perché escludere da questo tavolo anche Bin Laden e tutto il movimento di Al Qaeda? Le ragioni sottostanti, addotte da Fassino a giustificazione delle proprie affermazioni, a ben vedere, potrebbero anche adattarsi a questi ultimi. Noi auspichiamo al più presto una ritrattatazione da parte del Governo, signor vice Ministro, a nome dello stesso Fassino, già oggetto di numerose critiche a livello internazionale per questa proposta che offusca la lieta notizia della liberazione di Mastrogiacomo, critiche di cui il nostro Paese assolutamente non necessita. Pochi mesi di confusa e sconsiderata politica estera di questo Esecutivo, in una fase cruciale come quella che stiamo vivendo a livello internazionale, stanno cancellando anni di buone relazioni intessute ad arte dal precedente Governo. Non a caso proprio alla politica estera è collegata la prima e sicuramente non unica caduta di questo Governo che verrà per lo più ricordato per i continui e plateali scontri tra i suoi componenti, ultimo, ma solo in ordine di «apparizione», quello tra Prodi e il ministro Parisi, che ci fa dedurre che in realtà vi siano ben due Ministri della difesa: uno che manifesta preoccupazione, correttamente, per delle azioni che danneggiano una strategia posta in essere nell'ambito dei poteri del suo Dicastero, e un altro che, mettendo in atto strategie non concordate, ha ridicolizzato i nostri Servizi ma soprattutto mette in pericolo la sicurezza del nostro Paese. Ma ci chiediamo ancora se sia legittimo esporre così il nostro Paese a livello internazionale pur di accontentare e conseguentemente mettere a tacere le minacce della sinistra radicale. Non possiamo quindi non dedurre che Prodi preferisca soggiacere alle minacce dei terroristi talebani piuttosto che a quelle dei suoi alleati. Bisogna chiarire una volta per tutte se è opportuno o meno, ed è questo che infine chiedo, tanto al Governo quanto a quest'Aula, consentire la permanenza delle nostre truppe in Afghanistan, in Iraq, in Libano. I nostri ragazzi, da anni in questi martoriati Paesi, svolgono un ruolo di pace, di scolarizzazione dei bimbi afgani, liberano le schiave dai talebani, curano, anche attraverso le spedizioni con gli aerei della speranza in Italia, i giovani iracheni, ma nonostante ciò rischiano costantemente la loro vita senza poter contare su una nazione che riconosca il loro servizio, il loro sacrificio e il loro valore. Il Parlamento si deve finalmente esprimere, anche oggi in maniera convinta, senza tentennamenti, deve decidere attraverso il voto sulla permanenza delle nostre truppe nell'ambito di una linea strategico-politica, che questa è la verità, non è mai cambiata, soprattutto nell'interesse di quei ragazzi, dotandoli sia di adeguati strumenti di difesa che di assistenza. Fiori, opere di bene, ma anche la guardia alta quanto basta per salvare la vita, è un diritto dei nostri soldati, ed è un dovere di questo Parlamento.

Signor Presidente, desidero ringraziare innanzitutto il vice ministro Intini per la relazione ampia e dettagliata che ci ha proposto

Onorevoli colleghi, credo che il sollievo per la liberazione del nostro concittadino, giornalista de «la Repubblica», Daniele Mastrogiacomo ci accomuni tutti, insieme, naturalmente, al turbamento profondo per la barbara uccisione dell'autista e insieme alle preoccupazioni sulle sorti dell'interprete che accompagnava Mastrogiacomo nella sua missione giornalistica in Afghanistan. Credo che dovrebbe accomunare tutta l'Aula anche il riconoscimento che il Governo si è mosso nell'ambito dei limiti stabiliti da quella che ormai possiamo definire la tradizionale dottrina italiana in materia di sequestri di nostri concittadini all'estero. Una dottrina che distingue in maniera netta gli eventi di sequestro di persona con ricatto evidente, che si affermano in Italia sia ad opera della criminalità organizzata sia ad opera - in passato ne abbiamo avuto tragiche esperienze - di organizzazioni terroristiche, che non consentono il riconoscimento come interlocutori della criminalità o del terrorismo nel nostro Paese, dove vige e domina la legge italiana

e nel quale la dottrina italiana ha sempre posto come valore fondamentale da proteggere quello della vita e dell'incolumità dei nostri concittadini. Tale atteggiamento è stato seguito in maniera sistematica dall'attuale Governo e, negli anni scorsi, dai Governi che lo hanno preceduto. È stato seguito, in particolare, in circostanze ugualmente drammatiche, alcune delle quali risoltesi felicemente, altre meno, in Iraq negli anni scorsi. Unico limite invalicabile - che abbiamo sempre riconosciuto tutti come tale - è la non negoziabilità delle decisioni politiche del nostro Paese. Se il nostro Parlamento approva l'invio di una missione militare nell'ambito di istituzioni internazionali all'estero, tale decisione non è negoziabile sotto il ricatto del terrorismo. Ogni altro mezzo o strumento volto ad agevolare la salvaguardia e la tutela della vita dei nostri concittadini è stato esperito ad opera delle nostre forze di sicurezza, con il sostegno del Governi e delle opposizioni *pro tempore* in questa vicenda, come in quelle analoghe degli anni passati. Così come è sempre stato utilizzato - ove disponibile - il canale di organizzazioni non governative, umanitarie, che potessero essere considerate «terze» tra le parti e quindi agevolare il rilascio degli ostaggi. Non sempre questo atteggiamento e questa dottrina italiana sono stati compresi e accettati dai nostri alleati. Il caso drammatico che tutti ricordiamo è il caso Sgrena, che è ancora aperto per le sue conseguenze tragiche, una forma di contenzioso tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America. In questo caso, mi pare si possa affermare da chiari indizi quello che l'opinione pubblica ed anche noi abbiamo potuto cogliere, ciò che il Governo ci ha riferito oggi: pur non sempre condividendo, i nostri alleati hanno compreso; quindi, la difficile via della trattativa e del negoziato si è svolta senza determinare rotture nella solidarietà con i nostri alleati. Credo che la dottrina italiana su questo tema sia naturalmente discutibile, come ogni scelta di impostazione politica; tuttavia il fatto che sia stata sistematicamente seguita da entrambi gli schieramenti politici dimostra come essa sia profondamente radicata nella coscienza del nostro Paese e sia difficile

che sarebbero assolutamente ingiustificate; altra è la sede nella quale dovremo discutere, tra poche ore, della missione in Afghanistan. Questo è il momento nel quale riconoscerci nell'operato del nostro Governo riconoscerci nell'operato del nostro Governo e nella gioia per la notizia della liberazione del nostro concittadino, insieme - ripeto - al dolore, al cordoglio e anche all'orrore per la barbara uccisione del suo autista e alla preoccupazione per le sorti del suo interprete, rispetto alle quali chiediamo al nostro Governo di non lasciare nulla di intentato per favorirne la liberazione e la salvaguardia della vita.

Rivolgiamo un ringraziamento sincero a tutti coloro che hanno operato per raggiungere questo risultato. Esso è stato raggiunto anche perché il Paese ha dimostrato grande unità, come spesso succede quando vi sono passaggi difficili.Esprimiamo anche grande sdegno per la barbara esecuzione dell'autista: è nello stile dei terroristi disprezzare la vita e ricattare gli interlocutori. La vicenda, però, non è conclusa, signor Presidente. È incomprensibile l'arresto del capo del personale dell'ospedale di Emergency a Lashkargah, principale artefice della mediazione e del risultato raggiunto. non è ancora stato liberato l'interprete. Credo debba prevalere anche in questi momenti la diplomazia, la mediazione, la trattativa e la politica. Il ruolo di Emergency è stato determinante soprattutto a sud di Kabul, territorio nel quale il Governo di Karzai è debole o a volte assolutamente assente. È evidente che la trattativa non sarebbe stata possibile senza il consenso del Governo di Kabul e senza il consenso degli Stati Uniti: questo è innegabile! anche la dimostrazione, però, del nuovo ruolo della nostra politica estera, che dentro le alleanze internazionali riesce a garantire più autonomia, più autorevolezza, maggiore rispetto per i nostri alleati e maggiore rispetto per il nostro Paese. Paese. Deve prevalere la politica, anche per il futuro: noi vogliamo la conferenza di pace. Si sta polemizzando in questi giorni sull'eventuale presenza dei talebani a questa conferenza di pace: pace: si dice che è come se si sedesse allo stesso tavolo dei terroristi; oppure si polemizza sul fatto che questa proposta fosse finalizzata

I talebani, è innegabile, hanno conseguito due risultati: il riconoscimento politico e la liberazione di cinque prigionieri; questo non si può nascondere. Tuttavia, tutti i maggiori e più autorevoli osservatori internazionali ci fanno presente che è aperta da tempo una trattativa condotta dalla NATO con gli stessi talebani per il futuro di quell'area. Allora la NATO legittima i terroristi? Non scherziamo; è la politica che deve prevalere. Si sono liberati alcuni terroristi? Tuttavia la scommessa deve essere sempre quella di separare, attraverso la politica, quelli che sostengono il terrorismo da quelli che difendono il proprio territorio: questa deve essere la scommessa politica. È un azzardo? Però bisogna provarci; bisogna far prevalere la politica, costruire una posizione unitaria tra gli alleati per ottenere la pace; bisogna inoltre costruire un rapporto in quella regione coinvolgendo tutti i Paesi confinanti su un progetto di pace. di pace. Ripeto, è una scommessa, certo, ma bisogna provarci; forse è una scommessa, ma la politica deve prevalere perché l'intervento armato non ha prodotto i risultati che volevano essere conseguiti. Noi riteniamo che il Governo abbia operato bene, ma bisogna avere più fiducia anche nei confronti di coloro che avevano nel tempo denunciato i rischi della nostra presenza militare in quel territorio.

Signor Presidente, non si capisce perché, ma quando avvengono queste informative da parte del Governo su fatti importanti che toccano il Paese ci si carica di aspettative. Ahimè, per la mia breve vita parlamentare, devo dire che queste vengono sistematicamente deluse. Infatti, vice ministro Intini, apprezziamo la tempestività e la sua disponibilità a venire a relazionare

che tocca le persone, come anche casi personali che si intersecano con la vita politica e le vicende internazionali, non ci possono che vedere schierati schierati dalla parte di queste incolpevoli persone. Pertanto, chiusa la partita, anche noi siamo estremamente soddisfatti che la famiglia abbia potuto riavere

con i terroristi non si dovrebbe trattare; anzi, siamo sempre stati fermi su questa posizione. È possibile ora, o d'ora in poi, dare dignità di combattenti a dei terroristi? Perché questo sta accadendo, nel momento in cui trattiamo con queste persone. L'esito della vicenda per noi splendido: riavremo un giornalista che potrà scrivere in modo libero, su un giornale libero, in un Paese democratico; dall'altra parte, però, vi sono cinque talebani che non sono stati invitati ad andare in vacanza a vita, magari con una pensione pagata dagli organismi internazionali, ma si sa che, se poi hanno avuto anche moneta di riscatto, si riarmeranno, torneranno con i kalashnikov, ricompreranno tritolo, continueranno a tagliare nasi e orecchie ai loro connazionali che considerano dei collaborazionisti, e magari anche qualche altra testa

egregio Vice ministro, ma se l'operazione è stata condotta da Emergency, cioè da una persona, Gino Strada, lei mi deve spiegare:

accadrà prossimamente. Un giallo è stata questa vicenda, andata a buon fine, ma c'è stato anche un giallo nel giallo: il ministro degli affari esteri D'Alema

una parte dei colleghi della Casa delle Libertà, il collega Calderoli e il sottoscritto abbiamo presentato degli emendamenti perché le missioni militari all'estero si riducano non ad un anno, ma a sei mesi,

finanzia e si da continuità alle operazioni. È contraddicente con la volontà (o sedicente tale) di volere una pace subito. Vi è poi ancora qualche elemento a condire la vicenda: il segretario del Partito dei DS Fassino, che invita, o stimola ad invitare al tavolo addirittura i terroristi, i talebani.

perché se un'equazione molto semplice può essere questa: talebani significa integralisti islamici, gli integralisti islamici sono legati al sistema di Al Qaeda, Al Qaeda è la struttura responsabile

che gli americani, che vogliono chiuderla, questa partita, e vogliono arrivare a identificare e ad assicurare alla giustizia i responsabili di questa strage, possano sedersi, prima ancora di avere sconfitto Bin Laden, Al Qaeda ed i responsabili, ed accettino queste persone ad un tavolo di pace. È quantomeno velleitario pensarle, queste cose. Se si chiama qualcuno ad un tavolo di pace, significa che con i terroristi non si farà più guerra; è pensabile che gli americani, prima di aver avuto soddisfazione ed aver sconfitto tutto ciò che insidia il mondo occidentale, si possano sedere e far finta di chiudere una partita con queste associazioni? Un richiamo a noi: ma se noi avessimo avuto un attacco come quello che hanno subito gli americani, se avessimo avuto migliaia e migliaia di vittime civili, potremmo permetterci di sederci ad un tavolo con questi personaggi senza prima aver assicurato alla giustizia i veri responsabili? Lasciamo aperta tale questione, ma mi pare che le risposte da dare siano abbastanza semplici.

onestamente mi aspettavo qualche informazione in più; a differenza di qualche altro collega non ritengo che da parte sua vi sia stata una relazione abbondante e approfondita.

politica. In altri termini, intendo dire che la gioia umana riguarda il fatto, sul quale non vogliamo che ci siano dubbi da parte di nessuno, che la liberazione di una persona, in questo caso di un giornalista, ci sta particolarmente a cuore. Allora rivolgo una domanda, attraverso lei, al quotidiano «la Repubblica». Quando, nel corso del rapimento di Moro, quel quotidiano fu alla testa della linea della fermezza contro ogni ipotesi di trattativa, esprimeva una filosofia politica di fondo che fu definita, in una delle lettere di Moro, «ragion di stato».

Non si tratta di una continuità, di una politica trattativistica dell'Italia, ogni volta che vi è un rapimento di un italiano all'estero, come è stato detto. Occorre capire in quale contesto il rapimento è avvenuto e a quale trattativa si è dato luogo;

sapremo ancora una volta distinguere le nostre responsabilità internazionali, che sono per la continuità del nostro impegno internazionale continuità dell'impegno in Afghanistan, dovuta a una decisione internazionale assunta alla fine del 2001, dopo il gravissimo incidente delle Torri gemelle.

se questo tipo di rilascio, che è stato fondamentale, sia avvenuto prevalentemente per rapporti tra Governi, quello italiano e quello afghano, al di fuori di qualunque coinvolgimento delle nostre Forze armate. Vorremmo comprendere bene le ragioni per le quali non vi è stato nessun particolare apprezzamento per il Ministro della difesa. Vorremmo seriamente capire...

cogliere negli ultimi tempi. Ribadisco: gioia umana e forti perplessità politiche. Gioia umana perché la liberazione ci riguarda, ci ha riguardato sempre e ci riguarda anche in questo caso;

di disimpegno militare dell'Italia dall'Afghanistan? Vi è da parte del Governo l'idea della inutilità della nostra presenza militare? Se questo fosse l'orientamento, non potremmo, ovviamente, sostenere una missione internazionale che ha l'obiettivo opposto. Siamo per la continuità dell'impegno internazionale, non per la discontinuità, e lo siamo per ragioni esattamente opposte a quelle indicate da alcuni colleghi della cosiddetta sinistra radicale per essere stati favorevoli a questa trattativa. Non siamo contrari ad una conferenza internazionale,

ed è la seguente: quale diversa filosofia della politica il quotidiano «la Repubblica» esprime in ordine alle trattative che riguardano le persone sequestrate, avendo quel quotidiano posto la strategia della

Ed ha iniziato le trattative quando ha ritenuto di aver avuto la prova che la persona era ancora in vita. È il Governo italiano che si è mosso, non le Forze armate italiane. Questo è importante. Sono state informate di questa trattativa o ci siamo limitati a chiedere a inglesi e americani non condurre operazioni militari tali da suscitare opposizione nell'altro versante? I nostri sono stati determinanti nella trattativa o sono stati informati attraverso la stampa?

alla sostituzione delle Forze armate da parte di soggetti privati). Questo è molto importante, signor Vice ministro. Si tratta di disponibilità o di una sostituzione? L'ultimo punto. Il Governo afghano ha posto in essere degli atti formali (abbiamo sentito parlare di un decreto con il quale sono stati liberati i terroristi). È una forma di legittimazione internazionale o una forma di cedimento personale di Karzai? Lo abbiamo chiesto noi? Lo abbiamo sollecitato? Lo abbiamo, in qualche misura, indotto a fare questo? Lo abbiamo - per così dire - appreso? Qual è il grado di coinvolgimento italiano nell'azione del Governo afghano? Questo attiene alla natura della nostra presenza in Afghanistan. Ecco perché dico al collega Tonini che non vi è una sola generica continuità le trattative, ma una congiuntura specifica che riguarda l'Afghanistan, lo stato in cui oggi si svolge la missione e il futuro della missione medesima. Per questo ribadisco: gioia personale e forte perplessità politica. La gioia personale, ovviamente, è fortemente offuscata dal fatto che, delle altre persone,

dal ricordo di Sayed Agha, giovane autista afghano brutalmente assassinato dai talebani, e dal ferimento, fortunatamente lieve, di un nostro militare. Siamo felici perché sappiamo quanto sia dura una vita minacciata, tanto più dura in un contesto di guerra come quello. Questo esito politico ci parla comunque di una speranza, di una fiducia. Mi sembra che questa mattina il vice ministro Intini abbia ben interpretato tale sentimento e tale politica. Questo esito politico positivo è metafora infatti della speranza della fine di una guerra, cioè del contesto drammatico che ha portato alla grave situazione attuale. Emerge innanzi tutto un dato, che è centrale: Daniele è libero per un scambio, una trattativa, precisamente uno scambio di prigionieri; uno scandalo per gli ipocriti epigoni della linea della fermezza; ma *oportet ut* *scandala* *eveniant*, evangelicamente. Vi è invece finalmente una novità politica che viene dal lontano Afghanistan; sta appunto in quello scambio, nella trattativa, nel modo in cui si è realizzata. Ciò dimostra non solo che il negoziato non è precluso ma, anzi, che è il solo mezzo che garantisce risultati. Un negoziato molto ben condotto, che ha saputo coniugare la diplomazia ufficiale e quella del Governo, appoggiato da tutte le forze politiche, di maggioranza e opposizione, con quella stupenda risorsa, quel dono di comprensione e convivialità che è la diplomazia dal basso, il saper comunicare da popolo a popolo dentro la sofferenza; quella diplomazia che altrove è la cooperazione, come in America Latina, o il commercio equo solidale e le banche etiche delle donne, come in Africa, e che in quelle terre martoriate è costituita anche dai tre splendidi ospedali di Emergency di Gino Strada. Vedete, quel canale di trattativa e di testimonianza è possibile solo perché si pone al contempo dentro e contro la guerra, perché sta fuori dalle parti in conflitto, perché prende parte soltanto al fianco della gente mutilata dalle mine e dalle bombe, perché non chiede, quando vai a bussare alle porte di quegli ospedali, se sei terrorista o collaborazionista, ma ti considera una persona e quindi parla con te; quella persona parla con quell'italiano, con quegli ospedali. Questa è per tali motivi una voce ascoltata. È un dialogo che si riannoda, che parla contro la logica dell'*escalation* militare, che ci narra la povertà e la brutalità delle soluzioni e delle cornici militari, esclusivamente militari, e del tremendo ossimoro della guerra umanitaria. È un primo passo che ci dice dell'inizio della crisi della guerra preventiva globale, del ruolo importante di innovazione e di ricerca che questa maggioranza e questo Governo stanno svolgendo una difficile apertura di varchi di innovazione, di autonomia. È importante per noi che siamo una comunità, un gruppo pacifista, di un pacifismo non improvvisato, che ha conosciuto le sofferenze di Gaza come di Diyarbakir, come di tanti anni fa a Soweto o come quelle del 1994 nella Selva Lacandona e che quindi conosce la durezza e la pazienza della diplomazia dal basso e del pacifismo dei popoli, oltre ai gesti eclatanti e di coscienza. Noi siamo stati e siamo contro ogni guerra e siamo per l'unità articolata del movimento pacifista e non votiamo né voteremo mai i crediti di guerra. Vedete, se pensassimo anche solo per un momento che un nostro voto contrario al decreto sull'Afghanistan oggi in discussione riportasse anche un solo militare italiano a casa e alleviasse le sofferenze di quel popolo (che avverte la presenza militare, anche quella

che ci vuole imporre peraltro soltanto il Governo statunitense. Noi vogliamo resistere alle minacce di chi ci intima di permettere ai militari italiani di sparare, e di farlo sempre di più. Noi pensiamo sia possibile agire una riflessione comune e generale a livello internazionale e nazionale sui disastri delle guerre umanitarie; una riflessione che ci sembra l'unica strada realistica, l'unica strada politica (il realismo dell'utopia, diceva Bloch).

aperto una riflessione, che oggi il Governo sta portando avanti, su una iniziativa internazionale, una conferenza di pace, che già ora sta facendo discutere sconvolgendo gli schemi tradizionali bellici delle Cancellerie, mettendo in difficoltà lo stesso Governo statunitense (come l'incontro di ieri ha dimostrato), perché induce l'Europa, la Francia, la Germania, la Spagna ad uno schieramento positivo, perché parla di una soluzione politica, prendendo atto del fallimento dell'*escalation* militare. La liberazione di Daniele Mastrogiacomo ci incoraggia molto, ci dà fiducia, ci dice che è stata lanciata una manciata di sabbia negli ingranaggi di una guerra che sembrava inarrestabile, ne sono state fermate velocità e volano inerziali. Vi è una novità: si è creato un effetto di attrito. Forse è sul serio più vicina la soluzione politica per quanto riguarda l'Afghanistan. Le destre mi pare si scandalizzino o facciano finta di scandalizzarsi (ho sentito gli interventi di questa mattina) perché è stata posta la necessità di coinvolgere in qualche modo i talebani in senso politico, ovviamente - al tavolo delle trattative per la pace. Ebbene, vi sono al riguardo mille esempi, ma vorrei qui ricordare che le trattative fra NATO e talebani sono aperte da tempo, come sa chiunque si interessi di politica internazionale. Il presidente Karzai continuamente parla,

bolscevico filoterrorista, ma il generale De Gaulle, affermò, in uno dei suoi più famosi interventi che, se si vuole la pace, si parla ovviamente con coloro che sparano. Noi sappiamo che la conferenza internazionale non è dietro l'angolo e che non è obiettivo facile, ma il nostro auspicio è un impegno pressante, un impegno forte - noi vogliamo essere uno stimolo pacifista a questo impegno - che poniamo senza tregua al nostro Governo. Rifiutiamo il cinismo della *Realpolitik* (questo è il punto), che in qualche modo affida agli interessi del più forte, ad interessi di diplomazie internazionali, peraltro in crisi, la soluzione nel teatro afghano, perché non diventi un nuovo Iraq (ma sta diventando,

dall'Iran alla Siria, ovviamente alle forze della NATO, all'Europa come protagonista, ma anche - non dimentichiamole - alla Cina e all'India, che devono e possono svolgere un ruolo importantissimo. Se il Governo italiano riuscirà ad essere coagulo e stimolo di questa iniziativa, avrà fatto un'azione politica importante e noi appoggeremo fino in fondo l'azione politica del Governo italiano, che è l'unica che può portare, nella regione martoriata

Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio innanzitutto chiedere scusa al collega Russo Spena per averlo interrotto. Non è nel mio stile, però devo dire che il passaggio sul voto alla missione in Afghanistan

coalizione, di maggioranza e non certo un motivo di sentimento e di moto dell'anima, come tentava di venderlo il collega Russo Spena in quest'Aula. Devo dire al Governo che siamo profondamente insoddisfatti della sua presentazione e relazione perché - e non è la prima volta che lo diciamo - non è che le audizioni del Governo in Aula devono essere la raccolta delle agenzie ANSA. Queste le facciamo già noi da soli, non abbiamo bisogno che lo faccia l'ufficio stampa del Ministero; attendevamo qualche valutazione e giudizio. Non è vero che non è successo nulla; non è vero che le reazioni sul piano internazionale e per quanto riguarda la nostra politica estera siano così

La responsabilità che si è assunto chi ha avviato la trattativa era per tre persone, e non per una sola. Non è un caso che, mentre noi salutiamo oggi - certo con soddisfazione e gioia il rientro dell'italiano Daniele Mastrogiacomo, dobbiamo dire con grande franchezza che sentiamo pesante la responsabilità, come italiani, della morte di Sayed Agha, l'autista di Daniele Mastrogiacomo, e siamo estremamente preoccupati per la scomparsa di Ajmal Nashkabandi, l'interprete di Mastrogiacomo. Sono responsabilità politiche, sono responsabilità verso le famiglie, sono responsabilità soprattutto verso la comunità afghana che - voglio ricordare - ieri ha dimostrato contro la trattativa del Governo italiano davanti all'ospedale di Emergency, ritardando la partenza di Daniele Mastrogiacomo dallo stesso ospedale. La vicenda, quindi, come l'abbiamo costruita anche in Afghanistan, Karzai ha ceduto certamente alle pressioni del presidente Prodi, ma ha anche dichiarato che mai più loro afghani avrebbero liberato dei talebani in cambio di un prigioniero fatto dai talebani. Ciò vuol dire che abbiamo creato anche all'interno di questa realtà afghana una preoccupazione, abbiamo indebolito nell'immaginario collettivo la legittimità e la forza del Governo Karzai. Cinque anni fa le truppe dell'ONU

abbiamo indebolito Karzai e lo abbiamo fatto - lo ricordo al collega Russo Spena - ancor di più insistendo per la presenza dei talebani alla conferenza di pace. I talebani sono un problema afghano, sono un problema di Karzai, non sono un problema del Governo italiano. Il Governo italiano nella comunità internazionale riconosce legittimamente un solo rappresentante del popolo afghano: Karzai. È nell'autonomia del Governo afghano, è nell'autonomia del presidente Karzai decidere i metodi, le procedure, le possibilità o meno di colloqui con i talebani, come con tutte le altre componenti tribali e politiche. Non spetta a noi decidere quello che deve fare il Governo Karzai. Continuare a sostenerlo in tutte le sedi, continuare a sostenerlo in sede internazionale vuol dire indebolire e delegittimare un Governo per il quale noi abbiamo presenti 2.000 uomini sul territorio. Abbiamo costruito la debolezza dell'immagine degli italiani in Afghanistan. Oggi i talebani sanno che prendere un italiano significa poter recuperare quattro o cinque o sei - dipenderà dal numero di uomini - comandanti e portavoce che ritorneranno, come ha già fatto uno dei liberati, a invocare la *Jihad* e a comandare le truppe ribelli e terroriste dei talebani. Anche questo è un prezzo che pagheremo. Le preoccupazioni manifestate in tal senso dal Ministro della difesa sulla presenza degli italiani in Afghanistan dimostrano che questa operazione è stata condotta in maniera molto spregiudicata e non consona alle normali regole delle trattative internazionali. Vorremmo anche conoscere dal Governo le ragioni per le quali, essendo la provincia di Helmand sotto il controllo dell'*intelligence* britannica, di fronte alle dichiarazioni degli inglesi che erano pronti a condurre un'operazione militare con le forze della SAS il Governo italiano ha risposto pesantemente di no, nonostante le sollecitazioni del comando ISAF e quelle dei comandanti britannici. Anche questo certamente, specialmente se lo leghiamo al caso di Abu Omar, dimostra come oramai tra il Governo italiano, le istituzioni italiane e gli alleati e i *partner* dalla NATO vi sia un velo di diffidenza e certamente di non fiducia reciproca. Voglio parlare anche di questa benedetta diplomazia dei movimenti o diplomazia dal basso, come l'ho sentita chiamare questa mattina, invocata da Russo Spena e proclamata anche dal presidente della Camera Bertinotti. Mi pare che ogni tanto si scopra l'acqua calda, nel senso che forse qualcuno qui dimentica che, ad esempio, non più tardi di 15 anni fa, nel processo di pace del Monzambico che, credo, gli italiani con più orgoglio dovrebbero rivendicare (perché è l'unico processo di pace avvenuto in Africa sotto la nostra guida che ha ottenuto un risultato positivo),

né mai si contestò il ruolo e la guida della politica italiana, dei funzionari della diplomazia, del Governo italiano di allora e dell'allora ministro degli affari esteri Emilio Colombo. Quindi non è la prima volta. Certo, qualcuno deve saper stare al suo posto ed è questo l'aspetto grave. Credo che le dichiarazioni di ieri di Gino Strada siano da condannare, perché nessuno è stato autorizzato, a nome di non si sa chi, a criticare le azioni del Governo Karzai o addirittura ad accusare il presidente Karzai di aver messo i bastoni fra le ruote oppure a dichiarare che il presidente Karzai ci ha messo otto ore a liberare due afghani che erano a 500 metri della sua abitazione. Forse ad Emergency, forse a Gino Strada, che è certamente un grande chirurgo, occorrerebbe ricordare che la politica ha i suoi tempi, che non sono legati ai tempi della cultura di Emergency. Emergency. Inoltre, nel momento in cui si fa l'esaltazione di Emergency - e certamente va fatta - vorrei ricordare che in Afghanistan esistono molte altre organizzazioni non governative, molti altri operatori e volontari che offrono al popolo afghano la stessa assistenza, la stessa cultura, la stessa solidarietà di Emergency, che non è unica, non è sola e non ha il monopolio della solidarietà in nessuna parte del mondo. Credo che aver delegato aver delegato a Gino Strada (come risulta da parte del Governo), aver rinunciato alla politica in questa trattativa sia stato un altro grande atto di debolezza. Ne ha approfittato certamente Gino Strada, che avrà molti pregi: uno di questi è quello di essere molto bravo ad avere visibilità, perché il meccanismo di Emergency richiede anche, per mantenere il *brand*, un *marketing* molto attento e spinto. Non vorrei paragonare Gino Strada alla marchesa di Castiglione, ma nella storia del mondo ci sono state molte...

Oggi - mi avvio alla conclusione, signor Presidente - il problema che affronteremo nella discussione sul rinnovo delle missioni internazionali che la missione italiana in Afghanistan è profondamente diversa da quella che noi avevamo immaginato e costruito cinque anni fa e mantenuto per anni. Noi avevamo inviato una missione all'interno della NATO, operante nel quadro ISAF, con truppe che dovevano garantire la sicurezza; voglio ricordare che ancora ieri il ministro degli affari esteri D'Alema ha dichiarato che la sicurezza in Afghanistan è prioritario elemento per la stabilità del Governo Karzai, cercando di riportare questa missione a quella originaria. Oggi, soprattutto con le dichiarazioni emerse dalla maggioranza, abbiamo dubbi o quasi certezze che i nostri militari siano esposti in una missione estremamente pericolosa e dovremo essere molto chiari su quale deve essere il ruolo delle truppe italiane in Afghanistan. Oggi sono molto deboli all'interno dell'ISAF, molto isolate all'interno dello schieramento militare e sono purtroppo, nonostante quanto qui dichiarato, ormai in prima linea, se è vero come è vero, che i talebani della provincia di Helmand, attraverso il passo di Farah, stanno arrivando nella provincia di Herat, che è a noi assegnata. Quindi, è stata certamente una gioia rivedere ieri sera Daniele Mastrogiacomo, ma la politica ha altri tempi ed altri elementi e siamo estremamente preoccupati per il prezzo politico che pagheremo per questa operazione.

tutta l'opinione pubblica italiana ha vissuto in questi giorni. Credo però sia altrettanto corretto ringraziare anche le istituzioni che in maniera esemplare si sono adoperate per ottenere tale risultato. Parlo delle istituzioni che hanno lavorato all'ombra, quelle che non erano di fronte ai riflettori, quelle che non hanno cercato in tutti i modi di portare un loro rappresentante a marchiare un'operazione riuscita con il rilascio - e la soddisfazione per questo - del giornalista Mastrogiacomo. Mi riferisco all'unità di crisi della Farnesina, all'ambasciatore italiano a Kabul e a tutti i suoi funzionari. Vede, signor Vice ministro, al di là della sua scarsa attenzione, credo che... Rilevo che anche adesso sta ridendo con il suo collega. Probabilmente questo è l'atteggiamento che il Governo italiano ha nei confronti del dibattito Adesso se ne va perché probabilmente ha esaurito il suo compito.

quanto è successo e non quello che c'è scritto sui giornali. È un fatto grave, signor Vice ministro. É grave perché il suo è stato un intervento reticente, superficiale, un intervento che non ha dato alcuna risposta alle domande che addirittura non il Parlamento, ma i giornali

l'operazione che era stata in qualche modo già definita è stata poi annullata, creando una polemica con gli amici inglesi? E poi ancora il silenzio - come è stato chiamato - del ministro Parisi di fronte alle manifestazioni di soddisfazione espresse da tutti, che testimonia l'estromissione dei Servizi segreti del nostro Paese. Questo è un fatto molto grave, perché i Servizi segreti del nostro Paese,

costituiscono un elemento di grave debolezza per la sicurezza di tutti quanti noi. Questo è decisamente uno dei punti chiave sui quali avremmo avuto il piacere di sapere esattamente perché il *diktat* di Gino Strada - così come è stato ricordato da molti mezzi di informazione - è stato accettato dal ministro D'Alema, e quindi i Servizi italiani sono stati estromessi dall'operazione per il rilascio del nostro connazionale. Ma è stata anche innovata una procedura che voi chiamate «la diplomazia dei movimenti». A parte il fatto che il collega Mantica l'ha espresso con chiarezza, da sempre si utilizzano tutti gli strumenti possibili per operazioni come queste, ma non lo si fa in maniera sostitutiva, perché sono - per così dire - complementari, aggiuntivi. In questo caso, Gino Strada e la sua organizzazione si sono completamente sostituiti - da quello che dicono i giornali

avremmo avuto piacere di ricevere più dettagli, o meglio di ricevere dettagli, perché non ce n'è stato neanche uno e quindi è impossibile aggiungere qualcosa al niente. Ed ancora: quale è stato il costo politico di questa operazione? Il costo economico è certamente importante, ma tutti quanti potremmo anche condividere la necessità di essere solidali nei confronti di un connazionale in difficoltà. Penso che questo possa essere sostenuto da tutti, però il costo politico è altrettanto

i canali con i quali noi ci esponiamo a livello internazionale. Ed ancora, abbiamo preso in considerazione le dichiarazioni del mullah Dadullah, che dice: «Questa operazione ci è riuscita bene. Adesso siamo in grado di prendere qualche altro ostaggio, visto che questo ci consentirà di liberare i nostri connazionali dalle carceri»? Questo sta a significare che abbiamo indebolito non solo la nostra posizione in Afghanistan, ma anche quella di tutta la comunità internazionale; significa anche che le nostre truppe, sulle quali discuteremo quando

costituendo in Afghanistan. Questo scenario fa sì che sia assolutamente necessario sostenerle fino in fondo con equipaggiamenti adeguati alle nuove necessità.

per affrontare la battaglia di tutto l'Occidente contro il terrorismo. Come si fa a legittimare i terroristi quando il primo e più importante obiettivo della comunità internazionale è quello di chiudere questo capitolo vergognoso della nostra storia, che è il terrorismo internazionale? Questa operazione, alla fine, ci consente di dire che siamo contenti che sia stato liberato Mastrogiacomo, ci fa piacere sul piano della solidarietà umana e anche sul piano di una operazione che consente alla famiglia di riabbracciare il suo caro, ma sul piano politico il prezzo che abbiamo pagato e che pagheremo sarà molto, molto elevato e credo che il Governo italiano e il Parlamento

Presidente, non solo mi unisco alle espressioni dei colleghi e delle opposizioni in ordine alla soddisfazione e alla gioia per la liberazione di Daniele Mastrogiacomo, ma sono anche orgogliosa che il mio Paese difenda i suoi connazionali e sia in grado di operare per la loro liberazione. Mi chiedo quale sarebbe stato lo scenario della discussione di oggi se l'obiettivo che il Governo italiano, nelle sue istituzioni massime e con impegno pieno,

perché avviene oggi, colleghi. Infatti, lo scudo del dire di non aver aperto bocca durante le trattative trasforma le vostre posizioni di oggi non in un esercizio di politica, ma in un esercizio di strumentale polemica, e voglio adoperare questo termine perché è proprio delle Aule parlamentari e perché ho troppo rispetto per voi. Cominciamo con quelle che sono le prime valutazioni, le più comuni, tra quelle che sono state esposte. Il rapporto con i Governi degli Stati Uniti e della Gran Bretagna: mi pare che il vice ministro Intini abbia riferito compiutamente su questo e, se devo giudicare da quello che la stampa internazionale riferisce oggi in ordine alla presenza del ministro D'Alema, alla forza del suo discorso e al successo che ha riscosso nella comunità internazionale rispetto alla proposta della conferenza di pace, dovrei dire che quello che oggi avete affermato è privo di fondamento. Sono arrivate numerose critiche per quella che è stata ritenuta una sottovalutazione, o peggio, del ruolo dei nostri Servizi di sicurezza, in particolare del nostro Servizio militare per la sicurezza.

sottolineare la gravità di affermazioni rese dal presidente Berlusconi che riguardavano l'irrilevanza e la delegittimazione del ruolo del nostro Servizio per la sicurezza militare, proprio per dare il senso di quella che era la cifra del modo di stare al mondo della polemica politica in un momento in cui così grave era lo stato delle trattative. Non comprendo poi come non si possa cogliere la forza innovativa della conferenza di pace, così come il ministro D'Alema l'ha annunciata e proposta in sede ONU, e come su questo possano innestarsi polemiche che hanno piuttosto, ancora una volta, il carattere della strumentalità. Ma uno dei temi fondamentali che avete affrontato è stato quello del ruolo svolto da Emergency e da Gino Strada in questa vicenda. Devo allora ricordare il ruolo che svolse Scelli e la rivendicazione che fece del proprio, unico, ruolo nella liberazione delle due ragazze volontarie e anche le parole che pronunciò circa il fatto che il SISMI l'unica cosa che aveva fatto era aspettare all'aeroporto. Allora, colleghi, se vogliamo ragionare di politica e se qui oggi si è acceso un dibattito (ma anche ieri nelle trasmissioni televisive alle quali, per brani, ho assistito), emerge la questione se questo Paese debba porsi rispetto al sequestro di nostri connazionali

Contestualizziamo diversamente quello che fu il dibattito politico che assistette ai tragici fatti relativi al rapimento del presidente Moro,

polemiche politiche - che in questo Paese da anni ormai si tiene tanto alla vita dei nostri connazionali che si tratta; si tratta in cambio di denaro e si tratta in cambio di altri soggetti che sono l'oggetto della trattativa per il rilascio. È così. Allora discutiamo a carte scoperte, in condizioni di parità, perché nessuno può venire qui a innescare polemiche strumentali dimenticando il passato. Riteniamo che un Paese in questo contesto e in queste condizioni debba ragionare politicamente, non in termini di guerriglia politica,

Gruppi* *Ulivo e RC-SE)*, come lo fu durante i giorni del rapimento Moro. Questo è il punto politico. E se non siete in grado di affrontare politicamente questo

io: dopo la liberazione di Daniele Mastrogiacomo, dopo quello che sta accadendo in questi giorni all'ONU, questo tipo di atteggiamento riduce nell'ambito riduce nell'ambito stretto stretto della polemica contingente e strumentale un tema che invece è molto serio e rispetto al quale credo - se vogliamo - che dobbiamo confrontarci molto seriamente, sapendo che la verità di questi di questi anni è una verità non nascondibile, che il tema politico è gravissimo e che ciascuno di noi ha rispetto ad esso la stessa identica responsabilità.

Io ho predisposto una risoluzione rispetto a quanto comunicato nel dibattito; so che l'accordo è quello di non discutere o votare mozioni, ma proprio perché le questioni politiche sul campo sono così importanti

la ristrettezza dei tempi, chiedo la cortesia di poter consegnare il testo scritto, che riassumerò rapidamente.

n. 4 del 2007, recante proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali, in un clima - va detto - assolutamente costruttivo e dialogico. Nel voto finale in Commissione tutti i Gruppi si sono espressi a favore del decreto-legge con la sola significativa eccezione della Lega Nord

tutti i Gruppi, tranne la Lega Nord, hanno votato a favore del mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Aula. Tutti gli emendamenti presentati in Commissione sono stati respinti, anche se dalla maggioranza alcuni di essi erano condivisi nella lettera e altri, comunque, nello spirito. La ragione del parere contrario dei relatori e del Governo è stata il vincolo tecnico che, come è noto, impone che il decreto sia convertito entro i 60 giorni: il termine è prossimo alla scadenza e non ci sono i tempi tecnici per una terza lettura.

Come relatori abbiamo entrambi espresso l'impegno a raccogliere lo spirito di alcuni emendamenti in ordini del giorno e se ne parlerà nel momento opportuno. In questa breve relazione vorrei evidenziare tre importanti convergenze che hanno unito la discussione in Commissione.

apprezzamento per la loro professionalità, per il valore e per il senso di umanità che contraddistingue la presenza italiana in queste missioni internazionali. La seconda convergenza ugualmente importante è la precisa volontà espressa dalle Commissioni esteri e difesa di rafforzare i meccanismi di verifica parlamentare dei risultati delle missioni.

centro-sinistra. È una preoccupazione tipicamente parlamentare, cioè dell'istituto parlamentare, della sua funzione di controllo e verifica sull'operato del Governo. Noi intendiamo avviare un preciso programma di valutazione dell'efficacia, della congruità e dei risultati delle missioni, per ovviare ad un inconveniente che si è sistematicamente verificato in questi anni: quando si tratta di rinnovare le missioni, quindi attraverso decreti o disegni di legge di rinnovo del finanziamento alle missioni, la discussione e il dibattito si concentrano al massimo sulla missione che in quel momento crea più problemi dal punto di vista dell'opinione pubblica che quindi ha maggior visibilità nel dibattito pubblico. Finiscono sistematicamente nel cono d'ombra missioni che hanno uguale, se non maggior rilevanza in termini d'impegno di uomini e mezzi da parte del nostro Paese, che però non hanno la stessa visibilità visibilità politica. In particolare, è ormai da anni nel cono d'ombra la nostra presenza nei Balcani, che pure è una presenza straordinariamente significativa in termini quantitativi e che insiste in un'area nella quale si manifestano ancora focolai di tensione ed alcune grandi, irrisolte questioni politiche, come il futuro del Kosovo, che possono essere poi elemento di alimentazione di nuove tensioni e - speriamo di no - anche di nuovi conflitti. È quindi indispensabile avviare un percorso di valutazione sistematica di queste missioni, attraverso un programma di audizioni da parte delle Commissioni esteri e difesa del Senato nei confronti del Governo (Ministero degli affari esteri e Ministero della difesa *in primis*), per poter arrivare ad una valutazione la terza questione sulla quale si è concentrata la discussione è, ovviamente, la missione in questo momento politicamente più esposta e più problematica, cioè la missione in Afghanistan. Afghanistan. Nella valutazione su questa missione vi sono toni e sensibilità molto diverse nell'arco politico (questo è noto a tutti), divergenze di analisi sulla situazione di fatto e anche d'impostazione politica, tuttavia credo che innanzitutto vada valutato come un fatto politicamente rilevante che nessuna forza politica ha chiesto il rientro immediato dei nostri soldati dal teatro afghano, quindi c'è la consapevolezza che dobbiamo in qualche modo far fronte ad un dovere, ad una responsabilità che ci siamo assunti

innanzitutto una tendenza al peggioramento della situazione in Afghanistan, preoccupazione che ha unito tutte le forze politiche; la sicurezza e il controllo del territorio, la lotta al narcotraffico, la costruzione dello Stato, lo sviluppo economico, il progresso civile e culturale dell'Afghanistan restano obiettivi di non facile raggiungimento. La tendenza all'aggravamento è ulteriormente accentuata dall'instabilità dei Paesi confinanti, a cominciare dal Pakistan, che non vuole - o più probabilmente non può - controllare la sua lunga frontiera con l'Afghanistan, che si va trasformando in un'immensa zona franca per la guerriglia allo stesso tempo talibana, qaedista e del narcotraffico. Si è aperta, com'è noto, anche in conseguenza di questa difficile situazione, una discussione anche accesa sulla necessità di rafforzare l'impegno militare della NATO e, in particolare, di rivedere le regole d'ingaggio, più da *peace keeping* che da *peace enforcing*, adottate da alcuni Paesi europei tra i quali l'Italia (e insieme a noi la Germania, la Francia, la Spagna). In realtà, per quanto riguarda l'Italia, lo sforzo in termini di uomini e di mezzi è tutt'altro che modesto: con 2.000 soldati ed uno stanziamento di 310 milioni di euro, il nostro è uno dei contingenti più numerosi, il quarto praticamente a pari merito, per così dire, con la Germania - dopo Stati Uniti e Regno Unito. Il problema afghano è più ampio e più grave rispetto a quello di un rafforzamento della nostra presenza militare o di In Afghanistan c'erano all'inizio dell'inverno, schierati dalla NATO su mandato ONU, in tutto circa 36.000 uomini, uno ogni 25 chilometri, uno ogni 1.115 abitanti.

non può essere quella militare la soluzione al problema afgano, perché per rendere congrua la nostra presenza militare, ammesso che abbia senso questo ragionamento, dovremmo moltiplicare per dieci. I sovietici avevano 300.000 uomini e hanno perso la guerra. Per queste ragioni, la discussione si è sviluppata sulla dimensione politica del problema afgano e sulla proposta del Governo di una conferenza internazionale sull'Afghanistan, che il Governo è impegnato a promuovere in sede ONU, in Consiglio di Sicurezza. Ieri si è tenuta l'importante relazione del ministro D'Alema in Consiglio di Sicurezza, che ha riscosso primi incoraggianti segnali di attenzione da parte di grandi Paesi come la Germania, presidente di turno dell'Unione Europea, e degli stessi Stati Uniti d'America. Su tale punto si è concentrata la discussione e immagino che su di esso si svilupperà il nostro dibattito in quest'Aula. Signor Presidente, signori senatori, signori rappresentanti del Governo, rispetto alla...

il decreto di proroga, da oggi in Aula per la conversione, estende le autorizzazioni di spesa dalla cadenza semestrale a quella annuale e accentua, già nel titolo, la finalità umanitaria della partecipazione italiana alle missioni internazionali. In conformità al titolo, il primo articolo del disegno di legge dispone interventi di sostegno alle popolazioni dell'Afghanistan, del Libano e del Sudan e assegna un contributo all'Unione africana per l'istituzione della forza internazionale di pace in Somalia, deliberata dalle Nazioni Unite. Per l'Afghanistan, in particolare, a sostegno della popolazione è stato stanziato un finanziamento, finanziamento, elevato dalla Camera dei deputati dagli iniziali 30 milioni a 40 milioni, ed in parte destinato ad alimentare i fondi dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il contrasto alla produzione e al traffico di droga. Un finanziamento aggiuntivo è stato introdotto dalla Camera per l'auspicata Conferenza internazionale di pace per l'Afghanistan nell'ambito delle Nazioni Unite. Altri finanziamenti sono destinati a interventi di prima necessità, che siano disposti da contingenti militari italiani a soccorso delle popolazioni ancora in Afghanistan e, in misura minore, in Libano, in Kosovo e in Bosnia. Infine, il primo articolo autorizza la cessione gratuita di rilevatori di ordigni esplosivi per la bonifica del territorio libanese. Quanto all'Iraq, dopo il rientro del contingente militare italiano, l'impegno per la missione umanitaria di ricostruzione e stabilizzazione prosegue con gli stanziamenti autorizzati nel secondo articolo del disegno di legge, anche per la formazione e l'addestramento delle forze armate e della polizia irachene. Il terzo articolo proroga per il 2007 le missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, attive in tre Continenti, ma essenzialmente concentrate sui teatri operativi dei Balcani, dell'Afghanistan e, più recentemente, del Libano. Alle spese di indennità operativa di esercizio e di supporto logistico per le Forze armate dispiegate nei Balcani, in Libano e in Afghanistan è destinato oltre l'80 per cento dei 1.050 milioni stanziati dal disegno di legge. Il rapporto tra le finalità umanitarie e il carattere essenzialmente militare delle missioni è stato oggetto d'esame nelle Commissioni, in riferimento al fatto che di aiuti umanitari vi è nel mondo infinito bisogno anche in aree che non sono sotto i riflettori delle vertenze internazionali. E, in effetti, credo convenga riconoscere che quando le agenzie internazionali si determinano ad attivare a fini umanitari lo strumento militare, ciò risponde a situazioni in cui la tutela dei diritti umani ed il soccorso alle popolazioni locali si combinano con finalità ed interessi non meno legittimi, quali gli intenti di stabilizzare aree di crisi, prevenire o risolvere conflitti, contrastare il terrorismo nei luoghi della sua incubazione. Il titolo di legittimazione di ciò sta nella Carta delle Nazioni Unite, che autorizza l'impiego delle Forze armate contro le minacce o violazioni della pace e contro gli atti di aggressione ed è alla nascente organizzazione delle Nazioni Unite che pensavano i Costituenti italiani quando coniugarono, al ripudio della guerra, l'integrazione delle organizzazioni internazionali, nella prospettiva di un ordine di pace tutelata da istituzioni che abbiano il potere e gli strumenti necessari a garantirla o ristabilirla. Nell'esame delle Commissioni si è anche posta la questione della NATO in rapporto al quadro geopolitico del Trattato Nord Atlantico. Con la fine della Guerra fredda la storia non è finita. Sono insorte minacce di specie nuova, la cui novità consiste nella divaricazione fra la nozione di Stato e la nozione di nemico, nel senso che non sempre il potenziale nemico è individuabile in uno Stato sovrano. Dal 1999 l'Alleanza Atlantica ha, perciò, posto allo studio un nuovo concetto strategico che estende fuori area il concetto di sicurezza e di difesa, come è avvenuto dopo l'attacco dell'11 settembre 2001 contro le Twin Towers ed il Pentagono, con il ricorso all'articolo 5 del Trattato. Nel nuovo concetto strategico l'Alleanza atlantica tende ad accentuare l'aderenza con lo Statuto delle Nazioni Unite, già presente nel Trattato Nord Atlantico fin dal primo articolo, e a porsi direttamente al servizio delle Nazioni Unite; il banco di prova, dal 2003, è in Afghanistan con la Forza di assistenza per la sicurezza internazionale, affidata dal Consiglio di sicurezza al comando e al coordinamento della NATO. Il nuovo concetto strategico della NATO tende anche a sviluppare il partenariato con l'Unione Europea per rafforzarne reciprocamente le capacità, come stabilito nelle linee guida di lungo periodo definite nel Vertice atlantico di Riga. Dunque, le Nazioni Unite, l'Alleanza Atlantica, l'Unione Europea e la loro interazione sono le tre agenzie del multilateralismo in cui si inquadrano la politica estera italiana e la politica militare, che ne costituisce la proiezione necessaria. Al multilateralismo delle missioni internazionali l'Italia ha apportato in questi anni un contributo di primo piano segnatamente, sotto l'egida dell'ONU in Libano, dell'Unione Europea nei Balcani, della NATO su mandato dell'ONU in Afghanistan. L'esperienza acquisita nelle missioni internazionali ha trasformato la stessa concezione dello strumento militare, dalla visione statica della difesa nazionale affidata all'Esercito di leva, alla visione dinamica della sicurezza affidata a forze volontarie specializzate. Di fronte ad oneri, responsabilità e rischi che nessuno sottovaluta, si può affermare con certezza che le Forze armate italiane hanno dato nelle missioni internazionali prova costante - come ricordava poc'anzi il senatore Tonini - di alta professionalità, dedizione al dovere (fino al sacrificio) ed effettivo spirito umanitario verso le popolazioni vittime dei conflitti, sicché la loro opera - del resto sempre sostenuta da un largo consenso parlamentare - ha rinforzato il ruolo internazionale dell'Italia di fronte al mondo. Signori senatori, le 22 missioni autorizzate dal disegno di legge costituiscono la partecipazione italiana all'opzione del multilateralismo. Per riuscire efficace la via del multilateralismo presume l'interazione tra interventi politici, economici e militari e il ricorso allo strumento militare come proiezione di un mandato che deve commisurare i propri risultati al consenso delle popolazioni locali. Ed è alla stregua di quei risultati che devono essere valutati il mandato della partecipazione italiana alle missioni e la proporzione dei modi e dei mezzi predisposti per attuarlo. Nei lavori delle Commissioni l'adeguatezza delle forze e dei mezzi predisposti è stata posta in discussione in relazione all'aggravarsi della situazione in Afghanistan; se ne è sentita qualche eco preliminare già nella discussione precedente a questa. In Afghanistan l'interazione multilaterale è di piena evidenza, poiché la forza di intervento internazionale ISAF, cui l'Italia partecipa, deriva la sua legittimazione dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e delle Nazioni Unite, è stata dalle Nazioni Unite affidata al comando NATO e vede presenti la quasi totalità (per la precisione, credo, 25 su 27) degli Stati dell'Unione Europea. In quel contesto non si può affermare che al confronto con gli altri maggiori Paesi dell'Unione la partecipazione italiana sia di scarsa consistenza numerica. Dalla fine del 2005 ad oggi i contingenti di Germania, Spagna, Francia e Olanda risultano sostanzialmente stabili; quello della Gran Bretagna risulta ridotto, in attesa di rinforzi in arrivo fra aprile e maggio. Secondo i dati più recenti che ho potuto acquisire, la Germania è presente con 2.589 militari, la Spagna con 756, la la Francia con 1.036, l'Olanda con 1.469, la Gran Bretagna con 3.246, l'Italia con 2.117. Dunque, dopo la Gran Bretagna e la Germania, il contingente italiano risulta terzo tra gli europei per consistenza numerica. Quanto agli armamenti ed ai mezzi, vero è che le regole di ingaggio italiane si attengono al criterio della risposta proporzionata alle minacce prevedibili;

Le differenze che possono riscontrarsi fra l'armamento del contingente in Afghanistan e quello del contingente in Libano si spiegano per la differente configurazione delle minacce prevedibili: poiché in Afghanistan, a differenza del Libano, non sono prevedibili compiti di interposizione, non si è fatto ricorso ad armamenti quali i lanciamissili TOW ed i veicoli corazzati. Certamente nessuna valutazione in questa materia può mai essere definitiva e, qualora l'emergenza lo richiedesse, non mancano le pianificazioni e le procedure per incrementare le capacità. Signori senatori, è evidente che in Afghanistan non può esserci soluzione militare che non sia anzitutto e soprattutto soluzione politica; in quella direzione muove l'iniziativa italiana presso il Consiglio di Sicurezza per la Conferenza internazionale di pace, che dovrebbe riunire, insieme al Governo afgano ed ai Governi degli Stati confinanti, gli Stati che partecipano con impegno diretto, in rappresentanza della comunità internazionale, alla missione intesa a garantire finalmente condizioni accettabili di sicurezza e di stabilità al popolo afghano. La precondizione necessaria perché possa svilupparsi l'iniziativa italiana per la conferenza di pace è il mantenimento e la prosecuzione della missione in atto, che anche per questo motivo si raccomanda all'approvazione del Senato.

finestra") *(Ulivo)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quello di oggi è un passaggio veramente importante per la coerenza e la dignità del nostro Paese. Oggi siamo chiamati a decidere sulla proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali. Non c'è bisogno di ricordare quanto sia drammatica la situazione di quei Paesi e quanto siano necessari la nostra presenza e il nostro supporto militare e civile per la ricostruzione e per il ristabilimento della sicurezza e di condizioni di vita dignitose. Non credo che sia questo il punto di discussione. Come credo sia riduttivo, specialmente per l'Afghanistan, portare la questione sul dilemma guerra-pace. Siamo tutti d'accordo che il mondo sarebbe migliore se le armi non parlassero, se la politica fosse l'arma per eccellenza per risolvere i conflitti. D'altronde, la guerra non è più da tempo «totalizzante». La storia delle missioni militari italiane all'estero - dal Libano del 1982 all'Afghanistan - ha dimostrato che esiste ormai un «modello italiano», un approccio diverso al territorio e alla popolazione, che è diventato negli anni esempio anche per Forze armate di altri Paesi. È per questo che ai nostri militari va tutto il nostro apprezzamento per la loro elevata professionalità. Ed è in questo modo, con questa storia, che noi siamo in Afghanistan. Ci siamo nell'ambito di un mandato internazionale, che già di per sé rappresenta una grande vittoria rispetto all'unilateralismo statunitense, protagonista della guerra in Iraq. Dice il ministro D'Alema che la coerenza è un presupposto essenziale per una politica estera efficace. Vorrei qui ricordare il lungo e sofferto dibattito che ci fu durante la guerra in Iraq, in cui da più parti, in particolare da chi allora stava all'opposizione, si condannava l'atteggiamento unilaterale degli Stati Uniti e si invocava l'ingresso in campo delle istituzioni internazionali, Nazioni Unite, in primo luogo, perché soltanto in quel contesto era possibile prevedere un intervento sul campo. Si diceva, allora, che gli Stati Uniti erano visti come invasori e che soltanto una missione internazionale avrebbe garantito la necessaria credibilità e il consenso delle popolazioni. Dove sarebbe la nostra coerenza, la nostra credibilità, se ci tirassimo indietro da queste missioni internazionali? Certo non bisogna nascondersi la realtà. La situazione in Afghanistan è ad alto rischio; sul campo le cose sono diverse, più drammatiche, di come possono apparire a noi, qui, da lontano. Abbiamo vissuto giorni d'angoscia per la sorte dell'inviato di «la Repubblica» Daniele Mastrogiacomo, la cui liberazione e stata frutto di dialogo e di negoziato. Cosi sarà anche per la pace in Afghanistan: non sarà mai frutto delle armi e degli eserciti, ma del dialogo, della diplomazia, della solidarietà e della costante promozione di tutti i diritti umani per tutti. Non dobbiamo dimenticare che in Afghanistan c'è la fame: il 53 per cento della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà. I dati ufficiali ci raccontano che il 70 per cento della popolazione non ha un lavoro legale, il 60 per cento non dispone di energia elettrica e il 70 per cento della popolazione adulta non va oltre l'istruzione elementare. Il tasso di analfabetismo femminile supera l'85 per cento e il tasso di mortalità durante il parto è il secondo più elevato al mondo, con 1.700 morti ogni 100.000 gravidanze. Numeri da brivido, in uno scenario di conflitti, divisioni tribali, di mancanza di quel senso d'appartenenza ad una collettività che fa di un insieme di popoli una Nazione. Ma è proprio in quella direzione che stiamo lavorando e non siamo soli. Come affermato nella Conferenza dei 60 Paesi donatori, svoltasi a Londra nel 2006, le priorità sono uscire dalla prima fase post-bellica e avviare una seconda fase dedicata allo sviluppo economico e produttivo di quel Paese. Non c'è libertà e giustizia senza un livello minimo di vita garantito: se non spezziamo la catena dello sfruttamento e della povertà non avremo sicurezza. Certamente c'è molto ancora da fare, ma non si può neanche negare che dei risultati, importantissimi, sono stati raggiunti. L'altra sera mi è capitato di vedere in una trasmissione televisiva una parlamentare donna in collegamento da Kabul. Parlava a viso scoperto, ragionava di politica, di scenari, entrava nel dibattito con competenza e grande dignità. Credo che questo sia un grande risultato in un Paese come l'Afghanistan dove la donna, da sempre, ha vissuto in condizioni drammatiche di oppressione. E' importante lavorare su questo fronte, ed in tal senso abbiamo chiesto e ottenuto dalla Presidenza del Senato, come donne parlamentari, al di là dell'appartenenza politica, il patrocinio ed il sostegno finanziario per la costituzione di un gruppo permanente di contatto tra noi e le nostre colleghe afgane, nel Parlamento, nel Governo e nella società civile. E' questa la *ratio* dell'ordine del giorno sottoscritto dall'Unione, per il quale auspico e chiedo lo stesso unanime e condiviso sostegno delle senatrici dei Gruppi parlamentari dell'opposizione. Ora chiediamo anche al Governo un impegno affinché promuova e sostenga, anche attraverso un supporto logistico e diplomatico, la costituzione del gruppo di contatto permanente con le donne afgane.

Le donne possono fare molto per cambiare la mentalità e dare una scossa profonda ad equilibri tradizionali. Su questo credo siamo tutti d'accordo e lo abbiamo dimostrato come parlamentari, unite in questa positiva consapevolezza. In nome di quelle donne che stanno combattendo la loro battaglia per una vita migliore e dignitosa, una vita normale, credo sia giusto e coerente mantenere i nostri impegni per la ricostruzione sociale, economia e politica di quel Paese martoriato da guerre infinite. Quelle donne non possono essere lasciate, gli afghani non possono essere abbandonati.

vorrei innanzitutto esprimere la mia soddisfazione per il felice epilogo della vicenda Mastrogiacomo e ringraziare il Governo e tutte le forze, a partire da Emergency, che si sono impegnate nella liberazione del giornalista del Quanto all'Afghanistan, concordo con quanto dichiarato dal ministro D'Alema al Consiglio di sicurezza dell'ONU. È necessario battere la strada della Conferenza internazionale se si vuole portare la pace in un Paese devastato da decenni di guerra. Proprio in merito alla missione in Afghanistan intendo, in questa sede, focalizzare l'attenzione su un aspetto particolare, illustrando l'ordine del giorno a mia firma: l'Italia ha assunto una sfida decisiva, consistente nell'assunzione di un ruolo di guida per la ricostruzione del sistema giudiziario nel Paese. Tutto ciò avverrà unitamente alle autorità afghane e all'UNAMA. di *leading* *country*, ovvero di Paese guida per l'assistenza al Governo afghano nell'opera di ripristino di uno Stato di diritto, condizione essenziale per la nascita di una democrazia e, in particolare, per la ricostruzione di un'efficace amministrazione giudiziaria in grado di rispondere adeguatamente alla diffusa domanda di giustizia nel Paese, nel rispetto degli *standard* internazionali Il nostro Paese ha, dunque, il delicato compito di fornire un'assistenza tecnica qualificata al Governo di Kabul, nel rispetto della sua sovranità tentando la complessa conciliazione delle sue tradizioni della della *Sharia* con il rispetto dei trattati internazionali. Molti sono gli obiettivi già raggiunti. È utile, ad esempio, ricordare il contributo fondamentale prestato per la redazione del codice di procedura penale, del codice minorile e delle leggi penitenziarie. Molti altri obiettivi ancora restano da perseguire. Mi riferisco alla fondamentale riabilitazione delle istituzioni della giustizia, cioè del Ministero della giustizia e della Corte suprema e della Procura generale, alla formazione di giudici, procuratori, avvocati e quadri direttivi del Ministero della giustizia. Proprio in relazione a tali scopi, si vuole impegnare il Governo a valutare l'opportunità di predisporre adeguate risorse da destinare al rafforzamento istituzionale ed al sostegno all'amministrazione afghana nel settore giustizia attraverso l'invio *in loco* di magistrati e funzionari del Ministero della giustizia e l'organizzazione di corsi di formazione per magistrati e personale dell'amministrazione penitenziaria afghani a cura del Ministero della giustizia in Italia e in Afghanstan. *(Applausi della

Presidente, le missioni internazionali hanno visto la partecipazione dell'Italia per portare il proprio contributo al conseguimento delle condizioni di rappacificazione e per innescare un processo di sviluppo sociale ed economico; così è avvenuto ovunque: nei Balcani, in Afghanistan, in Libano e in Iraq. Questo si è verificato nell'ambito degli accordi con i Paesi alleati e nell'ambito degli impegni della comunità internazionale. Anche in Iraq, la recente Conferenza lascia sperare in un processo di rappacificazione. I contatti tra Stati Uniti, Iran e Siria sono segnali positivi, ma oggi siamo particolarmente preoccupati per la situazione in Afghanistan. L'intervento della comunità internazionale nell'ottobre 2001 è stato accolto dalla stragrande maggioranza degli afghani come una liberazione. Ce lo ricordavano i rappresentanti delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea in Afghanistan, in occasione di una recente audizione qui in Senato. Da allora, però, dobbiamo constatare, come hanno riferito gli stessi rappresentanti, che la comunità internazionale non ha aiutato a sufficienza l'Afghanistan. Ieri, il ministro degli affari D'Alema ha affermato che in Afghanistan noi possiamo e dobbiamo fare di più. E ancora, che ci sono stati significativi successi e che l'Italia è orgogliosa di avere contribuito al loro raggiungimento. Al tempo stesso, come sappiamo, è prevedibile un'offensiva talibana, e sempre il rappresentante delle Nazioni Unite esortava a non abbandonare la popolazione afgana ed esprimeva la preoccupazione della stragrande maggioranza del popolo afgano per l'eventuale ritorno al potere dei terroristi talebani. Sempre D'Alema ieri affermava che la guerriglia sta arrivando anche ad Herat e che non crede che le truppe italiane siano in una buona situazione. Quindi la situazione sta cambiando. Da qui la duplice preoccupazione: in primo luogo, che il Governo italiano non avrebbe ancora messo i nostri contingenti nella condizione di garantire una efficace difesa attiva; in secondo le recenti dichiarazioni del segretario DS circa la presenza dei terroristi talebani ad un futuro eventuale tavolo di una Conferenza per l'Afghanistan. Un riconoscimento, questo, politico, che dà forza ai terroristi talebani. Allora, il Governo e la sua maggioranza devono evitare, secondo me, posizioni come questa ed eventuali colpevoli disattenzioni nei confronti dei nostri contingenti. Sarebbero posizioni sconsiderate e irresponsabili se dettate da equilibri interni dell'attuale maggioranza. Chiedo pertanto che il Governo chiarisca questi punti, e che chiarisca bene la propria posizione. Per questi motivi così importanti e delicati, io avrei preferito qui anche la presenza del Ministro. Signor Presidente, vorrei spendere qualche parola per illustrare il mio ordine del giorno. Sappiamo che in Darfur ci sono stati almeno 300.000 civili ammazzati e ci sono due milioni di sfollati. Il recentissimo Rapporto speciale delle Nazioni Unite sulla condizione dei diritti umani accusa la comunità internazionale di insensibilità nei confronti di queste azioni criminali e sollecita la stessa comunità internazionale ad intervenire e ad agire rapidamente. Per questo chiedo che il Governo l'Italia siede nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite - faccia di tutto presso le Nazioni Unite e presso le sedi internazionali per fare in modo che in Darfur cessino le gravissime violazioni dei diritti umani. *(Applausi dal Gruppo FI.

Signor Presidente, signor Sottosegretario, il mio assenso al rifinanziamento della missione militare in Afghanistan nasce dalla persuasione che essa possa essere oggi, differentemente dal passato, uno strumento a sostegno della politica di pace condotta dal Governo italiano in quel contesto geopolitico, come del resto in altri, a partire da quello mediorientale. Ora, dunque, il problema è come garantire, coerentemente con l'articolo 11 della nostra Costituzione, che questa politica possa avere successo. La chiave di volta di tale politica in Afghanistan è la realizzazione di quella Conferenza internazionale proposta dal Governo italiano, inizialmente accolta con sferzante scetticismo, ora guardata con attenzione da altri attori sulla scena internazionale, non osteggiata dal Governo Karzai, non più esplicitamente rifiutata dagli Stati Uniti. Una tale Conferenza deve avere come principale obiettivo un processo di pacificazione interna - come è capitato anche a me di scrivere su «il manifesto» di circa un mese fa, e quindi al riparo di ogni sospetto di condizionamento scaturito dagli avvenimenti legati al rapimento di Daniele Mastrogiacomo - o, se si vuole, di riconciliazione nazionale, come ha detto il nostro Ministro degli affari esteri nel corso delle sue giornate all'ONU. Questo mi pare il senso dell'affermazione del segretario dei DS sulla possibilità di aprire anche ai talebani il tavolo di un eventuale negoziato di pace. Certo, per arrivare ad un tale risultato è necessaria una tregua e in questo quadro un mandato chiaro per le nostre truppe - che le metta in condizione di concorrere a realizzare un equilibrio anche militare tra le forze in campo, consapevoli come dovremmo essere che non ci sarà alcuna conferenza di pace se - da un lato - non si creano le condizioni politiche innanzitutto perché si fermi l'avanzata dei talebani, - dall'altro lato - non si mette fine alla guerra di annientamento di cui a volte sembrano tentate le truppe della NATO impegnate in prima linea in Afghanistan. Vorrei aggiungere che, prima che dal punto di vista politico, da quello culturale e storico appaiono infondate le analogie che vengono fatte da destra tra situazione afgana e vicenda del terrorismo italiano. D'altra parte, il fondamento tribale dell'assetto della società Pastun, su cui i talebani esercitano in particolare la loro influenza, ci debbono indurre a non fare valutazioni troppo semplici e indifferenziate sul fondamentalismo afgano e le sue potenziali articolazioni. Certo è che dopo l'11 settembre e lo scatenamento di «*Enduring freedom*» non si è fatto alcun passo in avanti nell'azione di isolamento dei terroristi di Al Qaeda, né tantomeno sono stati sconfitti i talebani, né risultato apprezzabile né risultato apprezzabile ha ottenuto l'azione della NATO. Voglio scommettere sulla possibilità di una svolta che riguardi l'Afghanistan ma anche nel suo complesso su questa epoca di guerra permanente che stiamo vivendo sul piano generale, e che per certi aspetti precede l'11 settembre e che inizia forse con la guerra nel Kosovo della fine degli anni '90. Mi piacerebbe che tutta la sinistra partecipasse a questa scommessa, senza defezioni, anche in nome della comune impresa che ci aspetta nelle settimane e nei mesi che verranno. Signor Presidente, signor Sottosegretario, signori senatori. Vorrei esporre alcuni dubbi e alcuni interrogativi - li esprimo a titolo personale - sulla missione in Afghanistan. È chiaro che ai nostri militari va tutto il mio personale sostegno e la mia stima per il servizio che sono chiamati a svolgere a favore della comunità internazionale. dobbiamo renderci conto che è cambiato il clima politico rispetto al Governo Berlusconi e che l'ambiguità dell'attuale Governo rende precaria, rende pericolosa la permanenza dei nostri uomini. Il compito del nostro contingente militare in Afghanistan è di promuovere e difendere i valori della libertà e della democrazia. Ma nel momento in cui è iniziata l'offensiva talebana mi chiedo: i nostri militari sono sufficientemente armati per rispondere a questo assedio - è di ieri soltanto la notizia di un attacco ai nostri soldati e del ferimento di un nostro soldato - o il Governo, per affermare un pacifismo ad oltranza invocato dalla sinistra massimalista, vieta loro di imboccare le armi? Come può essere credibile la nostra azione militare il cui obiettivo, sotto l'ombrello della NATO e dell'ONU, è quello di legittimare il Governo Karzai se le trattative per la liberazione di Mastrogiacomo - per fortuna a lieto fine hanno seguito il percorso inedito dello scambio di terroristi? È questa una modalità nuova che espone i nostri militari a futuri ricatti e che porta i talebani ad imboccare facili scorciatoie per ottenere vantaggi nella loro azione terroristica. E che dire poi della scelte di escludere il SISMI e il SISDE dal negoziato per affidarlo esclusivamente a Strada? E perché non è stato neppure consentito al SISMI la messa in sicurezza dell'ostaggio dopo la consegna ai volontari di Emergency? Che significato ha, da un punto di vista istituzionale, l'esclusione del Ministero della difesa a favore di un canale umanitario? È ancora una volta il movimentismo che prevale in questo Governo sul rigore delle istituzioni? E a che cosa si riferiva Prodi quando l'altro giorno, al telegiornale, ha ringraziato i Servizi segreti? Si riferiva forse ad un ringraziamento per la loro esclusione? Ma di più. Come fa il Governo a conciliare la nostra missione, volta al consolidamento delle forze democratiche, con l'invito ai talebani a sedere al tavolo della Conferenza di pace? Mastrogiacomo, nell'articolo sulla Repubblica che descrive la sua terribile e disumana prigionia, ha visto, nel comportamento dei talebani, l'odio verso chi, come lui, non è musulmano e anche la giustificazione della loro azione di combattimento nel trionfo dell'Islam. Mi chiedo: ma noi che cosa abbiamo da spartire con costoro, cosa abbiamo da spartire con gli autori del caos attuale, con i terroristi che hanno preparato l'attentato alle Torri gemelle. Cosa abbiamo da spartire con chi sgozza le presunte spie senza un processo? Non mi piace condividere nella politica estera l'irresponsabilità di Fassino e dei suoi compagni. Noi non potevamo, senatrice Finocchiaro, contestare un metodo da noi disapprovato finché Mastrogiacomo era ancora prigioniero e quindi mettendo a rischio la sua vita in Afghanistan. Non mi piace, dicevo, condividere la politica di chi mette sullo stesso piano quelli che difendono la libertà e la democrazia e quelli che invece ne minano le fondamenta: è come se noi considerassimo alla stessa stregua e invitassimo allo stesso tavolo i tutori dell'ordine e i mafiosi, i rappresentanti delle istituzioni e i brigatisti rossi. Io non posso assolutamente accettarlo. L'attuale Governo non fa questo per un'intima convinzione, peggio, lo fa per un meschino calcolo di bottega politica in un contesto di impossibili equilibrismi con la sinistra antagonista,

Da ultimo io non credo che la maggioranza e il Governo possano nascondere, dietro l'invito fatto all'opposizione ad una collaborazione sulla missione in Afghanistan, le loro incongruenze e le loro lacerazioni interne. Io non credo che questo Governo possa pensare che, allargando il numero dei voti parlamentari, da un lato aumenti il peso politico di una scelta e dall'altro vada a dissipare le perplessità del centro-sinistra. È tempo, e non è mai troppo tardi davvero, che questo Governo e questa classe politica si assumano le loro responsabilità di fronte agli elettori. È tempo che questo Governo, in mancanza di numeri, non cerchi legittimazioni esterne o comodi salvagenti per le sue decisioni. Mi auguro che la maggioranza conti su un'autosufficienza un'autosufficienza di 158 voti a suo tempo promessa al Capo dello Stato proprio sulla politica estera e non su altro. Non facciamo finta di ignorare che Prodi è caduto proprio su questo tema. Se ciò non accadesse, io credo che il Governo dovrà trarre le dovute conseguenze di un voto che indicherebbe politicamente la fine di una maggioranza in quanto tale. Certo non è un obbligo giuridico, ma morale e politico sì. Ne guadagnerebbero il senso di responsabilità, la coerenza, il rispetto della gente.

e 3-00498, presentata dai senatori Legnini e Ferrante, con le quali si chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministero intenda assumere relativamente alla scoperta, avvenuta a seguito delle indagini condotte dalla procura della Repubblica di Pescara per il tramite del Corpo forestale dello Stato, di una discarica abusiva di rifiuti tossici comprendente un'area di circa tre-quattro ettari in località Bussi (Pescara), a valle della confluenza del fiume Tirino con il fiume Pescara, sulla scorta di quanto comunicato dal Commissario delegato per l'emergenza socio-ambientale del bacino del fiume Aterno, dalla prefettura di Pescara, dalla Regione Abruzzo, dal Corpo forestale dello Stato, dal Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente e dall'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente (ARTA), si rappresenta quanto segue. La suddetta area, sita nelle immediate adiacenze dell'ex stabilimento Montedison, oggi di proprietà della Solvay, è stata ceduta nel 1999 dalla Montedison ad una società immobiliare di Milano e si trova a poca distanza dai parchi nazionali Maiella Morrone e Gran Sasso-Monti della Laga. A seguito dei sondaggi e carotaggi effettuati da tecnici di ditte specializzate e dal Corpo forestale dello Stato, con l'ausilio di geologi e chimici, sono state rinvenute, ad una profondità media di cinque-sei metri, sostanze tossiche e nocive, frammiste a terreni inquinati, riconducibili a idrocarburi clorurati alifatici come pentacloroetano e esacloroetano, impregnati di cloroformio e tetracloruro di carbonio che, per effetto delle piogge, cedono gli inquinanti al fiume. Le quantità stimate di materiali da rimuovere sono pari a 225.000-250.000 tonnellate, per un costo di smaltimento valutato in 57 milioni di euro. Credo si tratti di un fatto inaudito.

Al fine di accertare l'eventuale inquinamento delle falde acquifere, sono in corso, da parte del Corpo forestale dello Stato e dell'ARTA Abruzzo, indagini geognostiche nei terreni interessati mediante posizionamento di piezometri. Le risultanze delle analisi di laboratorio sui campioni di terreno e di acque prelevati verranno inviate alla procura della Repubblica e potranno essere utilizzate dall'ARTA per individuare l'entità e l'origine dell'inquinamento. Allo stato, la discarica è sottoposta a sequestro da parte dell'Autorità giudiziaria per l'accertamento delle responsabilità. Si potrebbero configurare i reati di disastro ambientale e avvelenamento delle acque. Il Commissario per l'emergenza del bacino del fiume Aterno, d'intesa con il procuratore della Repubblica di Pescara, ha convocato per il 27 marzo prossimo venturo una riunione del Comitato tecnico scientifico alla quale parteciperanno rappresentanti della direzione generale del Ministero che rappresento competente per materia e del Dipartimento della protezione civile. Già in quella sede, probabilmente, si potranno conoscere i risultati dell'indagine avviata dall'autorità giudiziaria. Nello stesso giorno è prevista anche una riunione presso la Prefettura e un sopralluogo nell'area in questione. Si sottolinea che all'esito degli accertamenti svolti dalla procura della Repubblica di Pescara, qualora venisse confermata una compromissione delle matrici ambientali, verranno assunte da parte del Ministero le opportune iniziative per il recupero del danno ambientale cagionato. In relazione, poi, alla richiesta del senatore Legnini di dichiarare lo stato di emergenza ambientale ai sensi della legge n. 225 del 1992, ovvero di attribuire al Commissario delegato per l'emergenza del bacino del fiume Aterno i necessari strumenti e risorse per fronteggiare la bonifica dell'area in questione, si fa presente che nel primo caso si rende necessaria la preventiva istanza della Regione, mentre nel secondo, al verificarsi di determinate condizioni e a seguito di intesa con la Regione, sarà possibile integrare l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3504 del 9 marzo 2006, richiamata nell'interrogazione. alla possibilità di classificare detta area quale sito di bonifica di interesse nazionale, si fa presente che tale qualificazione potrà avvenire a seguito della verifica dei requisiti e delle caratteristiche ambientali previste dalla normativa in materia

dell'immediatezza di questa risposta - le interrogazioni sono della settimana scorsa - anche grazie alla sensibilità della Presidenza del Senato che conosce questa situazione e, soprattutto, all'allarme che si è generato

strumenti, uomini e mezzi economici perché temo, purtroppo, che il problema sia di estrema rilevanza. Per quanto riguarda i provvedimenti successivi, sarà anche mia responsabilità e mio interesse associarmi insieme a tutti i colleghi abruzzesi per sollecitare le procedure che consentano di arrivare a interventi più incisivi e meglio strutturati.

ringraziare il sottosegretario Piatti e il Governo per la risposta tempestiva ed esaustiva; sono stati forniti tutti gli elementi che ci sono utili per farci ritenere che il fenomeno di cui stiamo discutendo è grave, grave, ha procurato allarme e impone interventi incisivi di una certa consistenza per fare in modo che il sito in questione venga bonificato al più presto. L'interesse della risposta del Governo relativamente ai punti che avevo posto con la mia interrogazione si palesa soprattutto relativamente agli strumenti che sarà utile attivare. per quanto ci ha detto il sottosegretario Piatti, non esclude l'utilizzo di nessuno degli strumenti previsti dal nostro ordinamento, cioè la dichiarazione di emergenza ambientale ai sensi della legge n. 225 del 1992, l'integrazione dei poteri, delle funzioni e dei compiti del Commissario delegato (che, pure, si è immediatamente attivato nei termini che abbiamo che abbiamo ascoltato); infine, la possibilità di classificare il sito in questione come un sito inquinato d'interesse nazionale. Questi strumenti potrebbero porre il Governo nelle condizioni di un intervento più efficace, di fornire dotazioni finanziarie nei modi e nell'entità che abbiamo ascoltato (si presumono cifre ingenti per poter provvedere al risanamento di questo sito); essi pongono quindi il Governo nella condizione di poter operare nel modo più efficace possibile. Continueremo a seguire, com'è doveroso che si faccia, questa vicenda per fare in modo che quel territorio e quelle popolazioni possano vedere risanato un sito industriale di interesse storico e d'interesse anche attuale, perché su quel Comune si stavano concentrando iniziative di grande interesse da parte della Provincia di Pescara, della Regione Abruzzo, degli enti locali, finalizzate a contrastare la deindustrializzazione e a sostenere la ripresa produttiva.

Presidente, nella seduta del 7 marzo ho sollecitato, ai sensi dell'articolo 153, comma 2, del nostro Regolamento,

La risposta non l'ho ancora ricevuta. Si tratta di un adempimento dovuto da parte del Ministro dell'interno, che avrebbe dovuto presentare al Parlamento un disegno di legge a seguito di un pronunciamento di sette Comuni della Valmerecchia, quindi della Regione Marche, che con *referendum* avevano in modo quasi plebiscitario chiesto di essere aggregati alla Regione Emilia-Romagna. Dopo quel *referendum*, il cui esito è stato regolarmente pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, il Ministro avrebbe dovuto, nei 60 giorni successivi, presentare al Parlamento il disegno di legge per dare attuazione a quel pronunciamento popolare. Il Ministro non l'ha fatto; sollecitato il 7 marzo non ha ancora risposto alla mia interrogazione, quindi mi trovo costretto a rinnovare la richiesta nella seduta odierna, nella speranza che il Ministro si decida non tanto a rispondere alla mia interrogazione, quanto a presentare il disegno di legge. Senatore Berselli, la Presidenza prende atto delle sue dichiarazioni. Provvederemo a sollecitare questa sua richiesta al Governo,